«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli dal 10 - emendamenti aggiuntivi - al 15, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 12.303, 13.301, 13.302, 13.303, 13.304, 13.305, 13.306, 13.307, 14.307 e 15.302. In ordine alla proposta 10.0.300 il parere è non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, al comma 1, all'inizio siano inserite le seguenti parole: "Per l'anno 2009"; che, al comma 1, dopo le parole "a tutela del consumatore", siano aggiunte le altre "per gli anni 2009‑2011"; che, al comma 6, la parola "quantificati", sia sostituita dalle altre "pari a". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 11.302 sulla quale l'espressione del parere è sospesa».

senatore Benedetti Valentini.

altri, intendono sopprimere le norme che in primo e in secondo grado, commi 3 e 5, andrebbero ad ampliare in maniera molto estesa, in maniera molto estesa, confusa e indeterminata la competenza delle così chiamate sezioni specializzate del marchio e del brevetto In verità, l'errore circa le competenze di queste sezioni è a monte, nelle precedenti legislature e sotto precedenti Governi di vario orientamento. Mentre le norme europee indicavano ai Paesi membri di istituire uno o pochissimi organi giudiziari del marchio e del brevetto con competenza esclusiva su queste precipue materie,

In questo modo, si è stravolto l'istituto, si sono sottratte competenze naturalissime a tutti i tribunali, grandi, piccoli e medi, diffusi sul territorio nazionale

inoltre, si è in contrasto con l'orientamento che abbiamo ormai adottato, cioè quello di eliminare il rito societario proprio per favorire la semplificazione

anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate», con un perimetro assolutamente indeterminato. Questa non può essere una norma che fa parte di una buona procedura. Per queste ragioni la Commissione giustizia, all'unanimità, ha approvato un parere che chiede, appunto, la soppressione dei commi 3 e 5 dell'articolo 11, lasciando quanto meno inalterata la situazione attuale,

quantomeno sulla soppressione dei commi 3 e 5, che riguardano il primo e il secondo grado, dell'articolo 11. *(PD)*. Signora Presidente, con l'emendamento 11.800 io ed i colleghi cofirmatari abbiamo ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sulla necessità di stabilire un collegamento tra il Consiglio nazionale anticontraffazione e organismi omologhi operanti nei Paesi esteri, sia nel settore della proprietà intellettuale ed industriale che nel settore della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari. Ciò al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto promossa, per l'appunto, dal Consiglio nazionale anticontraffazione.

conferisce funzioni di indirizzo, di impulso e di coordinamento delle azioni strategiche poste in essere da ogni amministrazione nella lotta alla contraffazione. Tutto questo al fine di migliorare e di condividere le conoscenze sulle azioni di contrasto alla contraffazione. Questa è sicuramente un'azione positiva, ma deve essere necessariamente accompagnata da quello che noi proponiamo... deve essere necessariamente accompagnata da quello che noi proponiamo in questo emendamento, e cioè che il Consiglio nazionale anticontraffazione debba ogni anno presentare al Parlamento una relazione sui risultati della lotta alla contraffazione nonché sull'attività svolta in quell'anno dal Consiglio stesso. Auspico davvero

possano essere partecipate anche dagli operatori che direttamente sono interessati alla lotta alla contraffazione.

non si dice nulla. Scusate, ma stiamo parlando di meccanismi giudiziari di una qualche delicatezza; ripeto, non sarà il cuore di questa legge che tutti sosteniamo e vogliamo portare all'approvazione,

che da parte del Governo e del relatore si spiegasse perché non possono essere accolti questi due innocui, semmai benefici, emendamenti. In caso contrario (non posso naturalmente costringere nessuno

Non vogliamo che per responsabilità che sono della maggioranza il senatore si permetta di inveire nei confronti del nostro Gruppo, attribuendogli responsabilità che, ripeto, sono tutte della sua maggioranza. Si cerchi altrove la responsabilità! Noi i nostri emendamenti li proponiamo, li difendiamo, cerchiamo di farli passare e abbiamo giustamente modificato in meglio questa norma.

11. 3 del senatore Maritati, membro della 2a Commissione. Ricordo molto rapidamente che questo emendamento fa riferimento alle norme in materia di competenza e, in particolare, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo

siamo convinti della necessità di sopprimere il comma 3 per motivi squisitamente tecnici, giuridici e processuali. Ne avevamo discusso ampiamente all'interno della Commissione giustizia, tanto che in data 4 marzo 2009 si era arrivati a un parere unanime in questo senso,

ed esplicitato durante i lavori della Commissione, anche in questa sede voteremo a favore dell'emendamento.

Il fatto che le Commissione giustizia, con approfondito esame e facendosi carico delle proprie competenze, abbia espresso un parere unanime significa che la Commissione competente, sia pure in sede consultiva, ha valutato tecnicamente lo stravolgimento determinato dall'estensione della competenza in questa materia.

Grazie,

contraffazione, poi c'è una inspiegabile opposizione ad un emendamento che tenta di salvaguardare il *made in Italy*. Le norme attualmente non sono affatto chiare e questo consente, per esempio, di fabbricare le scarpe in Cina, mettere le suole in Italia e poterci scrivere *made in Italy* se è stato fabbricato in Italia; oppure se in parte è fabbricato all'estero, però ha subito in Italia l'ultima trasformazione. Con l'emendamento 11.0.2, oltre a prevedere norme più stringenti per poter utilizzare il marchio, prevediamo che il manufatto italiano che riporta l'etichetta *made in Italy* debba indicare in apposita etichetta la filiera del processo di lavorazione e i Paesi che hanno partecipato alla sua realizzazione. È davvero inspiegabile

Il marchio *made in Italy* è uno dei più preziosi al mondo, perché deriva da una creatività e da una forte artigianalità nelle produzioni. almeno auspicare che vi sia una rintracciabilità della filiera produttiva vuol dire far emergere una enorme quantità di imprese che lavorano e partecipano ad un processo produttivo seguendo la regola d'arte, seguendo la perfezione del *made in Italy*. Mi rendo conto che fissare delle percentuali è sempre complesso. Purtuttavia abbiamo visto, signor Sottosegretario, in numerose circostanze marchiare con *made in Italy* o come prodotto puramente italiano delle produzioni, (anche di altissima gamma) che vengono realizzate per il 70, l'80 o il 90 per cento in Paesi nei quali non si rispetta nessuna regola contrattuale e nessuna clausola sociale, dove si utilizzano dei sottoprodotti e dove si utilizza anche il lavoro minorile. Io vorrei non solo apporre la mia firma e quella di tutti gli esponenti del Gruppo Partito Democratico in Commissione industria su questo emendamento, ma soprattutto sostenerlo davvero con spirito italiano, di salvaguardia delle produzioni italiane.

il *made in Italy* può essere posto su quei prodotti che siano realizzati in misura prevalente nel Paese.

Signor Presidente, prendiamo atto delle affermazioni del Sottosegretario.

non voglio far perdere tempo in alcun modo, né tanto meno mettermi in contrasto su un punto sul quale credo che abbiamo analoghi obiettivi.

Noi abbiamo sempre avuto grande difficoltà ‑ lei lo sa bene, perché ha seguito questi argomenti per anni - soprattutto per quanto riguarda il settore del tessile e dell'abbigliamento, a proteggere le nostre produzioni, anche a fronte di iniziative europee che, in fondo, hanno interesse a ridurre il valore aggiunto di questo marchio.

per la volontà di trovare delle soluzioni. Voglio anche ricordare che non più tardi del 1º maggio un'autorevole associazione agricola ‑ era presente anche il ministro Scajola ha svolto un'importante manifestazione per difendere la filiera italiana ed il *made in Italy*. Non voglio polemizzare sul fatto che l'Europa magari è quella dei banchieri e non quella dei cittadini,

possiamo accantonare l'emendamento, però voglio essere chiaro in quest'Aula. Non possiamo modificare le norme sull'etichettatura del Paese di origine,

È evidente a tutti che un prodotto fatto in Cina non può essere etichettato come *made in Italy*. Ove lo facesse incorrerebbe nel reato perseguibile come tale.

se non ci piacciono, dobbiamo modificarle in quella sede. La nostra battaglia dal 2003 è finalizzata a rendere obbligatoria l'etichettatura sul Paese d'origine nell'ambito europeo per i prodotti provenienti da fuori Europa. Ma questa battaglia passa attraverso un regolamento europeo

praticano una politica di difesa dei prodotti di qualità e dell'identità. Ricordo al riguardo la battaglia condotta ad Hong Kong, nel dicembre 2005, per la difesa delle indicazioni geografiche delle produzioni agricole non solo italiane, ma europee in generale. Quindi il nostro non è un atteggiamento nuovo. È un atteggiamento del quale siamo assolutamente convinti. È peraltro un atteggiamento che è stato spiegato nel modo più autorevole in occasione dell'Assemblea della Coldiretti la scorsa settimana dal presidente del Consiglio Berlusconi

più volte richiamato anche da interventi dell'opposizione, la Presidenza ha dichiarato inammissibili diversi articoli e commi del disegno di legge collegato nel testo proposto dalla Commissione. Dichiaro inoltre inammissibili, ai sensi della richiamata norma regolamentare, i seguenti emendamenti: 16.332, 16.333, 16.338,

così come sarebbe opportuno riflettere sull'ammissibilità dei commi 2*-bis* e 2*-ter* dello stesso articolo, Peraltro, sull'emendamento 12.302 è utile richiamare la circostanza che ha visto impegnata la Commissione

Quell'emendamento viene riproposto, seppure con l'aggiunta di un'autorevole firma, in questa sede, ma il testo è esattamente identico a quello ritirato in Commissione. Il provvedimento riguarda lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, e quindi le azioni tese a determinare condizioni di animazione del mercato al fine di suscitare un rafforzamento delle capacità competitive delle imprese e delle aziende operanti nei diversi settori e ciò al fine anche di rafforzare la capacità di penetrazione sui mercati internazionali. Queste norme, che ne modificano altre esistenti, vanno esattamente nella direzione opposta,

esplicito ed ufficiale pronunciamento dell'*Antitrust* attraverso l'espressione di un parere che è stato reso nelle forme definite dalle procedure relative all'attività della stessa Autorità. è disponibile, è all'attenzione di tutti noi e non merita ulteriori commenti. Per questi motivi chiedo di valutare l'ammissibilità di questo emendamento.

Le nuove compagnie che si affacciano sul mercato italiano (i Lloyd's in primo luogo) stanno aumentando a dismisura la raccolta e operano con il modello del plurimandato. Quello che non funziona in Italia, se vogliamo aiutare l'utente e l'assicuratore, è l'organizzazione. Abbiamo fatto una verifica cento dei dirigenti delle compagnie assicurative si trovano con due o più mandati in altre compagnie apparentemente in competizione.

sarebbe ancora condizionato dal monomandato, e ciò vorrebbe dire stravolgere ciò che di buono abbiamo ottenuto con la concorrenza, con l'apertura del mercato e con l'offerta plurima, sulla base sostanzialmente dei bisogni degli assicurati.

meno della metà. C'era il decreto Bersani, per offrire al mercato un minimo di concorrenza, e ora noi ritorniamo indietro.

finestra"). Se non vi sono altri interventi, vorrei manifestare il mio pensiero, che poi va a conferma di quanto già detto poc'anzi in occasione della dichiarazione di inammissibilità di altri emendamenti.

Grazie, Così abbiamo fatto e ci siamo adoperati in tal senso. La 5a Commissione è stata convocata *ad hoc*, per le valutazioni *ex* articolo 81 della Costituzione e per le dichiarazioni di inammissibilità. Questa Presidenza si è inoltre soffermata nel dichiarare alcune inammissibilità, testé formalizzate. Ritiene di non potere che confermare queste valutazioni rispetto ad altre che, invece, non sono state effettuate. Su questo punto, nel confermare l'ammissibilità del tema, mi permetto di segnalare ai colleghi che

secondo la Presidenza, il richiamo nel titolo alle parole «sviluppo delle imprese» contiene in sé, seppure in maniera astratta, la possibilità di intervenire nella disciplina dell'attività delle imprese, in quanto finalizzata,

sul giudizio di inammissibilità degli emendamenti, che ha anche adesso richiamato. Però ci permettiamo di insistere sulla

perché ogni settore del nostro sistema economico sarebbe astrattamente riconducibile alla materia dello sviluppo.

non parliamo di un provvedimento genericamente volto allo sviluppo dell'economia, ma dei temi, quelli dell'energia *in primis*, che sono contenuti nel testo originario e sottoposti al vaglio preliminare di ammissibilità nell'altro ramo del Parlamento, relativamente all'aderenza del contenuto stesso con la risoluzione la risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF. Non c'è alcun dubbio dal nostro punto di vista che la materia assicurativa è totalmente estranea sia al contenuto originario del disegno di legge, sia soprattutto al contenuto della risoluzione di approvazione del DPEF. del DPEF. Quindi, sia il comma 2-*bis* dell'articolo 12 sia l'emendamento a prima firma del presidente Gasparri,

che contenessero la clausola di esclusiva del mandato assicurativo. Qui si elimina questa parte importante,

Quindi, la invitiamo fortemente a rivalutare la sua decisione ed a dichiarare inammissibile sia il testo proposto approvato dalla Commissione sia l'emendamento 12.302.

non può rendersi protagonista di una violazione così palese del nostro Regolamento, forzandolo in modo inaccettabile ed introducendo una

Non voglio entrare nel merito perché lo abbiamo fatto già in Commissione e i colleghi conoscono perfettamente la posizione della Commissione, tant'è vero che sull'emendamento 12.300 si esprime contrarietà, perché la Commissione ha avuto modo

Sul tema dell'ammissibilità vorrei associarmi a quanto ha testé espresso il Presidente del Senato, perché definire il tema delle assicurazioni come un corpo estraneo rispetto al sostegno e allo sviluppo delle imprese mi sembra un po' improprio. Non vorremmo fare l'elenco degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, che probabilmente non rientravano specificamente

Noi parliamo dello sviluppo e della internazionalizzazione delle imprese e poi andiamo a restringere i margini di competizione in favore dei consumatori, ripristinando il sistema dell'esclusiva nel rapporto con gli agenti

in votazione, non potremmo che essere d'accordo con i colleghi della Lega e votare contro la sua approvazione.

in linea del tutto astratta, rimango convinto del fatto che in questo testo si possa affrontare la materia assicurativa, in quanto si tratta di sviluppo di un settore imprenditoriale o aziendale. Abbiamo espunto dal testo tante altre materie, a conferma del fatto che quando abbiamo trovato la motivazione e la fondatezza dell'inammissibilità ci siamo assunti le relative responsabilità. Si è dato luogo a un dibattito articolato e, siccome è intenzione ed interesse della Presidenza fare in modo che i lavori d'Aula e il confronto tra maggioranza e opposizione possano continuare su questo binario,

Grazie,

Grazie, Presidente. sul settore delle vendite a distanza, che in Italia presenta volumi nettamente inferiori alla media europea. Ciò a seguito del decreto legislativo n. 196 del 2003, che prevede la definizione di un codice di deontologia mai attivato. Considerato, quindi, che non si è ancora provveduto in merito e che l'intero mercato delle vendite è bloccato agli indirizzari del 2005, con grave danno non solo per il

Grazie,

ingannevole la pubblicità delle tariffe al netto di tasse e altri oneri aggiuntivi o comunque riferite a singole tratte di andata o ritorno.

non oggettivamente, ma soltanto tramite adeguamento con voci accessorie, come, ad esempio, la voce adeguamento carburante o diritti portuali. Sono quindi oneri accessori che si aggiungono al prezzo, alla tariffa, che non sono pubblicizzati. Chiedo pertanto che questo emendamento venga accolto proprio per favorire la pubblicità, l'informazione trasparente in favore dei consumatori e degli utenti del trasporto marittimo.

«Art. 12-*bis*. *(Introduzione dell'articolo 25-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime).* 1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: «Art. 25-*bis*. - *(Pubblicità delle tariffe marittime)*. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano, direttamente e in *code-sharing*, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte questi voci».

Chiediamo la verifica del numero legale.

Presidente, il Partito Democratico voterà contro l'emendamento 12.0.4, che propone una deroga al codice in materia di trattamento di dati personali con lo scopo di consentire invii postali finalizzati alla vendita diretta, al *marketing* e alla comunicazione commerciale. Non solo s'intende consentire l'invasione della vita privata dei cittadini italiani da parte delle rete commerciali di vendita o dei partiti o di qualsiasi altro soggetto, ma addirittura s'intende consentire l'utilizzo di generalità, di indirizzi dei destinatari, comunque raccolti, anche sotto forma di elenchi già esistenti. Chiunque pertanto sia in possesso di *mailing list* non utilizzabili per scopi commerciali perché costituite, per esempio, allo scopo di offrire un servizio, in questo modo potrà venderle senza che l'interessato ne sia a conoscenza ed anche se l'interessato nel fornire le proprie generalità ha firmato per un utilizzo limitato delle proprie generalità. Per questo, il Partito Democratico vota contro

la democrazia è garantita anche dalla pluralità dell'informazione. Questo è un convincimento sul quale il legislatore si è trovato unanimemente concorde sin da quando nel 1993 approvava la legge n. 422, che all'articolo 10 disponeva che una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione

era stato adottato sulla base di un precedente ordine del giorno, anche questo unanimemente approvato in sede di discussione alla Camera, nel quale si prendeva atto atto della stretta correlazione tra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese, con un esplicito riferimento agli aspetti inerenti la pubblicità. Orbene, voglio osservare che i suddetti finanziamenti non sono stati erogati all'emittenza privata nella modalità e nella misura previste dalla citata legge n 422 del 1993. L'emendamento 13.300 è finalizzato appunto a ristabilire questo disposto normativo, tenuto conto, tra l'altro ‑ questo vale la pena ricordarlo ‑ che l'emittenza televisiva locale rappresenta la prima forza lavoro del settore televisivo privato con oltre 5.000 dipendenti e l'effetto di ricaduta dell'attività dell'emittenza privata garantisce non soltanto i livelli di pluralità dell'informazione ma naturalmente rappresenta lo strumento sul quale si appoggia in modo solido il sistema di promozione e di pubblicizzazione delle produzioni locali, dei marchi dei territori e quindi del *made in Italy*. Auspico che tanto il relatore quanto il Governo vogliano trovare non soltanto gli elementi di coerenza contenuti in questo emendamento con quanto disposto dalla legge n. 422 del 1993, ma vogliano tenere conto

del nostro territorio in una logica di promozione anche delle specificità territoriali oltre che per gli aspetti attinenti la pluralità dell'informazione.

invito il senatore D'Ambrosio Lettieri a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Vi è una contrarietà del Governo addirittura sull'ordine del giorno, perché pare che tocchi l'aumento del canone, per cui non ci sono spazi per trovare motivazioni che possano indurmi all'accantonamento. Lo farei con piacere.

Grazie,

poche settimane fa è stato sostenuto da altro rappresentante del Governo nell'altro ramo del Parlamento, laddove su questi aspetti si è assunta la concreta disponibilità a verificare la materia dei finanziamenti delle televisioni locali in coerenza con quanto prevedono le disposizioni

per il 2010. Tutti ci rendiamo conto della difficoltà di una compatibilità finanziaria con la garanzia di questo principio rispetto alla situazione economica del Paese. Tuttavia, assumere un impegno sarebbe un segno di attenzione che interpreta non soltanto il disposto normativo, ma consente anche di restituire qualche spazio di speranza alla programmazione che l'emittenza privata fa nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda.

su tale argomento si dibatte spesso sia in quest'Aula che alla Camera dei deputati. Il Governo, come lei sa, ha recuperato il taglio che era stato effettuato sul 2009 recuperando 40 milioni che sono stati caricati sul 2008. Ora si parla di un ulteriore incremento. Il problema è che l'unico emendamento dichiarato ammissibile è questo proprio perché si vanno a prendere le risorse dal canone. Prelevare le risorse dal canone in questo caso ‑ lo dice l'emendamento stesso ‑ significa che, per determinare l'invarianza delle risorse per il servizio pubblico, si dovrà incrementare ulteriormente il canone a carico di tutti i cittadini.

del passaggio dall'analogico al digitale. Il che vuol dire che tutta l'emittenza locale, secondo uno schema di calendario determinato dal Ministero, avrà il vantaggio di avere non solo le erogazioni che sono già state previste precedentemente (e che vorrebbero essere aumentate in questa sede), ma anche tutto quello che le viene concesso in termini di comunicazione. Parliamo di decine di milioni di euro, che forse sono di più di quelli che si vorrebbero introdurre con questo emendamento. Quindi il mondo dall'emittenza locale riceve una grande attenzione

da dove le risorse vengono prelevate - una tale trasformazione mi sembra quindi complessa - ma, se per caso l'ordine del giorno dovesse mantenere il senso delle parole contenute in questo emendamento, fin da questo momento esprimo parere contrario.

tende a sanare un'antica ingiustizia. La legge n. 422 del 1993, frutto di un ordine del giorno unitario delle Camere, si dà all'emittenza locale la quota parte del canone che non va alla RAI. Il canone ha una quota percentuale che non va alla RAI, ma ad altre amministrazioni. Dunque le emittenti locali, sorrette da un voto unanime delle Camere di diversi anni fa, riuscirono a convincere il legislatore a promuovere una legge (la legge n. 422 del 1993) che in uno degli articoli recava esattamente questo punto che ora viene rievocato Quindi non c'è un aggravio, non c'è una sottrazione alla RAI: c'è semplicemente una piccola quota che comunque non va alla RAI, che comunque non farà aumentare il canone, che va ad altre amministrazioni e che dovrebbe andare, secondo una legge della Repubblica, all'emittenza locale. Ecco perché il tema è di grande delicatezza: si tratta di un'ingiustizia da sanare.

In ogni circostanza cui mi è capitato in diversi ruoli di assistere, si è sempre arrivati alla fine ad un ordine del giorno, che è rimasto sempre tale.

vorrei ringraziare il Governo per la sua disponibilità che, ancorché rappresentata

Cerchiamo di applicare al meglio il Regolamento, a garanzia di tutti. Vi è stata una richiesta di aggiunta di firme da parte di alcuni colleghi di opposizione al suo emendamento.

Grazie, conosciuto prima l'epilogo di questa vicenda e la posizione del Governo, non avrei avuto difficoltà. Ma poiché in questo momento il Governo, sia pure con toni generici, è disponibile ad accettare un ordine del giorno, non posso accettare l'aggiunta delle firme. *(Vivaci commenti

che con tanta virulenza tradisce il senso del garbo istituzionale, dimentica qual è la posizione politica che deve mantenersi anche in coerenza con la posizione del Governo e l'esigenza di raggiungere un obiettivo, credo che non soltanto offenda me - e questo mi rammarica - ma soprattutto mi duole che offende le istituzioni e l'Aula nella quale discutiamo.

È una delle possibilità che si possono dare nel caso in cui un emendamento presentato da un collega nel corso della discussione incontri il favore di altri senatori, i quali aderiscono alla proposta emendativa e aggiungono la firma. Ciò significa che nel caso in cui l'emendamento venga ritirato

Presidente, al di là del merito della vicenda in questione, a mio modo di vedere sembra porsi un problema che riguarda anche il futuro dei nostri lavori.

Quest'ultimo attribuisce al presentatore dell'emendamento una facoltà che egli deve esercitare preliminarmente, prima dell'inizio della discussione e di chiedere la votazione, prima che si svolga l'attività di cui all'articolo 102.

quando è intervenuto la prima volta, avesse detto di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno; tuttavia, questa facoltà non gli può essere più attribuita quando altri senatori, nella specie quelli del nostro Gruppo, hanno fatto proprio l'emendamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 102. Se passasse il suo orientamento, signor Presidente, si perverrebbe a un'interpretazione abrogativa dell'ultimo comma dell'articolo 102, perché è evidente che il presentatore dell'emendamento potrebbe in ogni caso neutralizzare l'esercizio della facoltà da parte dei senatori di fare proprio l'emendamento. Per

si determinerebbe la sostanziale eliminazione della possibilità per i senatori di far proprio un emendamento e questo non lo possiamo accettare.

altre sottoscrizioni. Ciò non era ancora avvenuto ed è prassi consolidata la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, che non comporta il ritiro dell'emendamento, ma la trasformazione e l'impossibilità conseguente che esso venga fatto proprio

Presidente, intervengo per chiederle di sottoporre la questione

emendamento venga considerata accettata se, immediatamente dopo essere stata avanzata, il primo firmatario dell'emendamento non dichiara immediatamente di rifiutare le firme che si propone di aggiungere. Nel caso che stiamo esaminando, il primo firmatario, nel momento in cui è stata avanzata da parte di alcuni senatori del Gruppo del Partito Democratico la richiesta di aggiungere le proprie firme, non ha

diversi, in tutti questi casi le firme in quel momento vengono considerate aggiunte all'emendamento di cui si tratta. Qui abbiamo avuto una *consecutio temporum* diversa, perché, dopo quello dopo quello che a mio avviso è stato un comportamento da parte del primo firmatario chiaramente di accettazione delle firme, è intervenuta un'altra fase

dobbiamo stabilire se, nel silenzio del primo firmatario, si configura l'istituto del silenzio-assenso, cioè l'assenso implicito, o se invece, in presenza di una richiesta di firma da parte di un senatore di una coalizione diversa, occorra l'assenso esplicito. Questo aspetto va disciplinato. Lei lo richiede, innovando la nostra prassi, e io sono d'accordo con lei sul fatto che la chiarezza non è mai troppa nei casi che danno luogo ad un dibattito d'Aula che ci sta impegnando da circa un'ora. Dunque, se è necessario

del Regolamento va a tutela del Parlamento perché, nel momento in cui c'è pressione del Governo sul parlamentare che presenta l'emendamento,

Lei sa meglio di me che spesso il Governo può spingere, forzare la volontà del presentatore dell'emendamento, che lo ritira malvolentieri. Questo è un punto importante nei rapporti fra Governo e Parlamento. Difendere le prerogative del Parlamento significa dare la possibilità agli altri senatori, nel caso ritengano che quell'emendamento contenga una proposta valida, di farla porre in votazione. La questione non è semplicemente formale

citando la prassi: ma può la prassi mettere nel nulla una disposizione esplicitamente prevista nel Regolamento? Ecco perché, signor Presidente, io la sollecito su questa questione. Del resto, non è la prima volta che, in quest'Aula, il presentatore di un emendamento finisce per votare contro il suo stesso emendamento: abbiamo assistito più volte passaggio, non certo esaltante.

Presidente, mi sono stupito del parere contrario perché in Commissione bilancio su quest'argomento vi era grande disponibilità sia della maggioranza sia del Governo. Mi stupisce perché questo emendamento fa risparmiare

dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento che - sicuramente non sarà sfuggito al relatore - ripropone sostanzialmente una serie di punti fondamentali attraverso una delega al Governo per migliorare e rafforzare il processo di liberalizzazione nel settore dell'energia, in particolare elettrica e - sottolineo - del gas. Questo provvedimento al nostro esame, infatti, come tutti hanno potuto verificare, è abbastanza complesso: tratta molti argomenti, e i titoli non rispecchiano esattamente i suoi contenuti. in materia di energia, si limita a riaprire la finestra sul nucleare, ignorando completamente o trattando in maniera molto frammentaria tutti quegli altri aspetti che riguardano il processo di liberalizzazione del mercato sia elettrico che del gas. Se l'Assemblea approva questo emendamento, viceversa, noi affidiamo al Governo un mandato, una delega perché fra l'altro possa legiferare e migliorare per esempio in materia di accordi fra gli Stati dell'Unione europea sulla sicurezza e l'affidabilità delle reti, sul tema delle compensazioni territoriali e - questo è un argomento che ha fatto molto discutere - sulla separazione societaria e proprietaria delle reti di trasporto del gas.

l'ENI debba uscire dalla proprietà della rete del gas fino al limite massimo del 20 per cento attraverso modalità e discipline che debbono essere stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Purtroppo in quella norma non è mai stato scritto entro quando questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere adottato: quindi, siamo

se venisse approvato l'emendamento 13.0.1, consentirebbe al Governo di operare è quello relativo all'introduzione di criteri di maggiore concorrenza nell'approvvigionamento del gas per quanto riguarda le forniture dall'estero. Confido quindi in un voto favorevole dell'Assemblea. *(Applausi